mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Vernetti. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro.

Al senatore Giannni Vernetti che cessa di far parte della nostra Assemblea, nella convinzione di interpretare anche il sentimento di tutti i colleghi, rivolgo un cordiale saluto e i migliori auguri di buon lavoro. Per consentire alla Giunta delle elezioni di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore dimissionario,

n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Puglia, a seguito dell'opzione del senatore Luigi ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Lorenzo

è stato il lavoro della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni ha deciso quanto ha appena letto il Presidente all'Assemblea, ma tutto questo è troppo criptico. Occorre aggiungere che, per il Regolamento della Giunta delle elezioni, per la Regione Piemonte il relatore ero io;

Ed era diversa perché io ritengo che non vi sia alcuna norma che consenta la possibilità di esercitare un'opzione postuma a chi, in effetti, è già senatore. Il senatore Bobba in questo momento, teoricamente, è senatore della Regione Puglia e senatore della Regione Piemonte. Tutto questo nessuna legge e nemmeno le norme più larghe previste dal Regolamento della Camera lo consentono. Ecco perché, rispondendo ad una logica nella quale non c'è un diritto privatistico sull'attribuzione del seggio, ma un interesse generale che nasce dall'indicazione degli elettori, e l'indicazione degli elettori per la Regione Piemonte prevedeva che dopo il senatore Vernetti che si è dimesso e il senatore Luigi Bobba che è stato già eletto in Puglia venisse proclamato eletto senatore il dottor Renato Cambursano, questa è stata la proposta corretta dal mio punto di vista

potrà essere corretta solamente dalla mannaia della Corte costituzionale, che dovrà purtroppo decidere che un potere di autodeterminazione può spettare ad un Parlamento serio, purtroppo, signor Presidente, non può competere ad un Senato come questo.

La mia breve osservazione sarà esclusivamente di carattere formale. Non entro nel merito di alcuna valutazione di tipo politico e ancor meno queste mie considerazioni investono le persone.

quindi, la decisione è inappellabile, contemporaneamente so però che avverso e contro le decisioni della Giunta medesima non il Senato della Repubblica, ma singoli senatori possono presentare ricorso. Io penso, signor Presidente, colleghe e colleghi, che non possa essere proclamata due volte una persona che già fa parte di un Parlamento. Ora, di fatto, la decisione della Giunta proclama eletto un senatore che è già eletto. È una cosa che è contro il buon senso, oltre che contro - spiegherò - la lettera e lo spirito della Costituzione repubblicana. Infatti, il Senato è eletto su base regionale; noi rappresentiamo un collegio regionale, una Regione, e riceviamo il mandato parlamentare su base regionale.

Non è possibile, quindi, che in una legislatura un senatore rappresenti per un certo periodo una Regione e per un altro periodo un'altra Regione.

per cui per un anno rappresenta il Piemonte, per un altro l'Emilia-Romagna, per un altro ancora l'Umbria, per un altro la Basilicata e per un altro la Sicilia. È evidente che è una condizione - certo soltanto ipotetica, ma che può diventare reale reale - del tutto inconsistente; tra l'altro, con una decisione di questo tipo, che viene assunta dalla maggioranza che si forma nel Senato, nel momento in cui tale maggioranza stabilisce di accogliere le dimissioni di un senatore, si contraddice totalmente - come ha giustamente detto poc'anzi il senatore Manzione - il mandato popolare, quello ricevuto dalle elettrici e dagli elettori, che viene contraddetto da una maggioranza parlamentare (in questo caso del Senato) che, arbitrariamente, decide chi deve essere senatore e chi non lo deve essere. *(Applausi dal Gruppo cioè ciascuno di noi, è già stato proclamato eletto in una Regione: questo vale per me, come per lei, signor Presidente, e come per ciascuno di noi. Il Senato, allora, a mio giudizio, non può assumere nessuna decisione, non può cioè esprimere alcun voto se non nel suo *plenum*. In questo preciso ad una situazione paradossale: c'è un senatore che vale per due. Questo non è possibile, non è formalmente accettabile. Per queste ragioni

A sostegno della tesi che invece la decisione sia corretta, si fa riferimento a precedenti che riguarderebbero la Camera dei deputati, che però, cari colleghe e colleghi, a differenza del Senato, non è eletta su base regionale. E qui sta la palese violazione della lettera e dello spirito della Costituzione nella decisione assunta dalla Giunta delle elezioni. La strada semplice, corretta e rispettosa della prassi parlamentare e costituzionale era quella di proclamare eletto il senatore che veniva nell'ordine successivamente e immediatamente dopo quel senatore di cui abbiamo accettato le dimissioni. Questa era la decisione semplice che la Giunta delle elezioni avrebbe dovuto assumere, prendendo atto che quello immediatamente successivo era già senatore della Repubblica e sedeva in quest'Aula. La decisione presa, pertanto, signor Presidente, cari colleghi, è - a mio giudizio - non conforme - lo ripeto - alla lettera e allo spirito della Costituzione, del Regolamento, della prassi e - se mi permettete - anche del buonsenso.

una considerazione diversa e la rivolgo a tutti i colleghi. Riguardo ciò che è avvenuto e ciò che potrà avvenire nelle successive votazioni, l'impressione che ho avuto, Presidente, è che noi abbiamo votato le dimissioni di un collega come se avessimo disbrigato un affare corrente (votazioni di un calendario, prolungamento dell'orario di una seduta e così via) e non abbiamo ben riflettuto su che cosa sta accadendo e su che cosa questo comporta. Penso che abbiamo compiuto un errore, indipendentemente dal collega che si è dimesso e indipendentemente dagli altri che lo seguiranno.

Non possono, a mio avviso, colleghi, dimettersi con motivazioni di carattere politico, quando queste motivazioni abbiano come contenuto quello di compiacere oggi il Governo, domani un partito politico, dopodomani un Gruppo o una corrente di un Gruppo. Il senatore ha uno *status*, un ruolo di gran lunga superiore che non può essere negoziato con nessun altro elemento di carattere politico. Credo che abbiamo mancato di riguardo

ci si dimette, si negozia, si guarda chi è il successore, si guarda qual è il vantaggio politico. Ma questo è il Senato della Repubblica, un organo costituzionale fondamentale, l'organo che preesiste e che sussiste prima e dopo la caduta di qualunque Governo! Noi abbiamo fatto tutto questo come se fosse cosa normale, ma facendolo abbiamo diminuito il prestigio e la funzione costituzionale del Senato. Io desidererei che questo non accadesse più e perciò, indipendentemente da coloro che hanno già presentato la domanda di dimissioni o da coloro che la presenteranno, quando le motivazioni siano di carattere politico, come queste, il Senato non accetti le dimissioni dei nostri colleghi per non mancare di riguardo alla funzione parlamentare. In caso contrario, io prego tutti i colleghi

che nella discussione della Giunta era evidente una consociazione di cui ho provato vergogna.

non lo so, ma sarebbe grave. So, però, che stiamo perpetrando un arbitrio.

della successione del senatore dimesso per le motivazioni che qui, con grande lucidità e forza politica, ha ricordato il senatore Angius.

e non la rappresentanza del voto popolare di un senatore proclamato, eletto e in piena carica. Per questo, io penso che ci sia stata una consociazione

deve tener conto, soprattutto per rivendicare l'orgoglio di quest'Assemblea. Abbiamo fatto tutti molto in campagna elettorale - non è retorica la mia

tutti coloro che hanno rassegnato le dimissioni di ritirarle e di far sì che venga meno questa sceneggiata e questa mancanza di rispetto nei confronti dell'Aula del Senato.

che, se ho inteso bene, si sono fermate un attimo prima di procedere alla definitiva proclamazione.

se dopo un anno e tre mesi optasse - sulla base di una scelta che io giudico, mi perdonino i colleghi, del tutto sciagurata, compiuta dalla maggioranza nella Giunta delle elezioni

vedete, non credo ci sia persona di buonsenso che non solo non veda cos'è avvenuto e cosa provocherà - lo dico anche assumendo, per quanto mi riguarda, la mia responsabilità - una violazione di questo tipo.

per uno scherzo, ma fu voluta dai nostri Padri costituenti esattamente per distinguere le basi e i mandati elettorali delle due Camere rappresentative del nostro Paese.

che oggi noi decideremmo che la Puglia è rappresentata in questo Parlamento da un senatore in meno, oggi decideremmo che ci possono essere atti che sono stati votati dal senatore Bobba in quanto senatore della Puglia

con il senatore Bobba che rappresenta un'altra Regione, altrettanto importante ma per la quale non era stato eletto in prima istanza.

l'abolizione della possibilità di candidarsi in diverse liste e in diverse Regioni. Lo dico tanto a coloro che sono contrari che a coloro che sono favorevoli: è chiaro che una decisione di questo tipo spianerebbe un'autostrada per che sostiene che quella condizione è insostenibile.

se un partito decidesse di presentare i medesimi candidati in tutte le Regioni fondamentalmente violerebbe la base, il recinto che la Costituzione prevede per la base regionale dell'elezione del Senato. Di fatto, si violerebbe uno dei princìpi fondamentali della differenza tra le due Camere e quindi l'elezione del Senato avverrebbe tranquillamente come quella della Camera dei deputati. Compiere un atto di questo tipo, quindi, provoca una lesione. Non si dica, se si va avanti,

perché personalmente ritengo che le decisioni della Giunta delle elezioni debbano essere accolte per quel che sono, ovviamente, criticate da chi non le condivide; con gli strumenti che ci sono offerti, possiamo naturalmente opporci alla loro esecutività. Io rispetto le decisioni della Giunta,

Il Governo, che ha la maggioranza nel Parlamento, ha ritenuto - e io condivido questa linea - che vi sia la necessità che i parlamentari dedichino il loro tempo al Parlamento e che i membri del Governo possano disporre di tutto il tempo che serve loro per esercitare le funzioni di Governo. in Aula il senatore Giaretta, che si è dimesso dal Governo per svolgere le funzioni di senatore; abbiamo altri senatori, membri del Governo, che si sono dimessi dal Senato dal Senato per poter svolgere le loro funzioni di Sottosegretari. Francamente, debbo dirvi che parlare di di costrizione da parte del Governo mi sembra assolutamente improprio.

negativo. Vorrei chiedervi - e lo chiedo a me per primo - quanti di voi hanno optato per più collegi e quanti di voi sono stati candidati in più collegi.

specificatamente su questo punto, che consideriamo particolarmente negativo, soprattutto per la funzionalità del Senato. La seconda considerazione che vorrei svolgere riguarda, invece, una contestazione politica grave che è stata fatta e che ho sentito ripetere proprio in quest'Aula. È stato detto, cioè, che la decisione della Giunta

non vi è stata mai non dico una trattativa, non dico un accordo, non dico una concertazione, ma nemmeno una una pressione; non vi è stato mai alcun tentativo nemmeno di condizionare il voto della Giunta. Quindi, amici, possiamo discutere di questo tema, com'è stato fatto legittimamente e con argomentazioni anche importanti, che dobbiamo prendere

questioni che non attengono al tema, perché qui non vi è stata alcuna trattativa politica e non vi è stato alcun inciucio. Così come non vi è stato certamente da parte del Governo né da parte della maggioranza alcun tentativo di costringere alcun parlamentare, che oggi siede nei banchi del Governo, a dimettersi dal Senato.

che alcuni colleghi abbiano accusato la Giunta, nella sua decisione, di aver agito contro la Costituzione, come ha fatto prima il collega Bordon. Dico soltanto che ha ragione ha ragione e straragione il presidente Pera nel dire che l'Assemblea sta affrontando la questione delle dimissioni con estrema superficialità.

Allora, Presidente, da membro della Giunta che ha assunto questa decisione e che si è sentito leso nella sua libera decisione, che non è stata contrattata con nessuno, chiedo a tutti colleghi di essere più rispettosi innanzitutto del loro ruolo e che le contraddizioni della maggioranza e del suo Governo non trascinino il Senato verso la perdita di prestigio e di credibilità. BUCCICO

i due blocchi, con il sopravvenire del sistema maggioritario la Giunta troppo facilmente si presta a votazioni o di maggioranza o, addirittura, di baratto tra maggioranza e opposizione; ipotesi che non voglio naturalmente insinuare, ma che si presta

del Piemonte e, giustamente, è stato ricordato l'articolo della Costituzione che prevede, a differenza della Camera, che le elezioni del Senato siano regionali.

Signor Presidente, non volevo intervenire in questa discussione per alcuni motivi. In primo luogo, perchè non sono uno specialista della materia, che evidentemente dal punto di vista tecnico è molto complicata e quindi va lasciata lasciata agli specialisti. In secondo luogo, perchè sono estremamente rispettoso delle decisioni della Giunta e tutti noi dovremmo esserlo perché, come è stato correttamente ricordato, nel Regolamento del Senato le decisioni della Giunta sono inappellabili. Quindi, l'Aula non può fare altro, a mio avviso, che prendere atto di quanto la Giunta ha deciso con un voto che reputo assolutamente regolare. Quindi, lascio le dietrologie a chi le ha fatte. Ho ascoltato, però, con grande interesse, gli interventi, anche di elevato livello, pronunciati in quest'Aula. Si è creato, colleghi, il classico caso di scuola, che spesso viene esaminato soprattutto in materia di legge elettorale o anche in materia costituzionale,

Quindi, ripeto, non avrei motivo per intervenire, se non per l'intervento del senatore Zanda, che normalmente argomenta in maniera molto pacata, ma che questa volta ha detto cose, almeno a mio parere (mi scusi, senatore Zanda), assolutamente inaccettabili perchè non è possibile, in un dibattito di questa natura, che si era tenuto su toni assolutamente elevati, introdurre la solita tiritera della legge elettorale. Tutta la colpa sarebbe della legge elettorale.

ce ne sono state molte in Italia e ce ne sono ancora di vigenti. Pensiamo, ad esempio, alla legge per il Parlamento europeo. Quindi, non buttiamo la croce addosso a questa legge per quanto è accaduto; soprattutto, senatore Zanda, non è colpa della legge elettorale se non avete avuto la maggioranza. Per governare ci vogliono i voti,

non per colpa della legge elettorale, ma perché godevamo di un vasto consenso elettorale. Questo è il dato fondamentale. Allora, per favore, prendete una decisione una volta per tutte. Non costringete il Parlamento a queste discussioni e a queste prese di posizione che derivano

avverso questa decisione, un senso di lacerazione del diritto e dell'estetica. Ecco perché ho interrotto - e me ne scuso - il senatore Stracquadanio mentre parlava. parlava. È vero che vi è l'autodichia e l'insindacabilità della decisione della Giunta, ma quando una decisione urta così violentemente il senso comune e il diritto è giusto e necessario reagire. Questa sera noi stiamo commettendo un delitto contro il diritto e contro il senso comune, nel senso che già questa Assemblea è costituita in questo momento in maniera irregolare perché il senatore Bobba si è sdoppiato in una doppia figura e rappresenta due senatori, snaturando la composizione elettiva di questa stessa Secondo il mio modesto apprezzamento, abbiamo vissuto una pagina non seria della vita parlamentare. Sotto questo profilo, mi permetto di dissentire completamente,

In conseguenza dell'opzione esercitata dal senatore Bobba per la Regione Piemonte, invito la Giunta delle elezioni a riunirsi immediatamente nell'adiacente Sala Pannini al fine di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore Luigi Bobba per la Regione Puglia. Sospendo pertanto

del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Puglia, a seguito dell'opzione del senatore Luigi Bobba per la proclamazione nella Regione Piemonte, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Lorenzo Emilio Ria.

ma non posso ammettere che, consultati gli organi e le persone istituzionalmente preposti a fornire risposte, mi si dica da una parte sì e dall'altra no.

vorrei chiarire le ragioni per le quali siamo favorevoli alla proposta di rinvio. Intanto, perchè ci piacerebbe avere il Presidente del Senato con noi: sicuramente importanti impegni istituzionali gli hanno impedito di partecipare ad una seduta in cui il relatore della Giunta delle elezioni ha dichiarato che, a suo avviso, la decisione assunta vìola la Costituzione, e altri autorevoli parlamentari, fra cui il Vice presidente del Senato, hanno ribadito tale opinione. Ci piacerebbe quindi avere il conforto del Presidente del Senato, ma questo pomeriggio non è fra noi. La seconda considerazione che voglio fare è che il senatore Zanda ha dichiarato che non c'è stato nessun accordo e il senatore Zanda è un uomo d'onore. Pertanto, è del tutto casuale che sulle dimissioni del sottosegretario Vernetti ci siano stati abbondanti voti in più rispetto a quelli della maggioranza per accoglierle ed è del tutto casuale che alla Giunta delle elezioni - ho sentito i nobili e ispirati interventi del presidente Matteoli e del presidente Pera - tutti i Gruppi del centro‑destra, compattamente, su una questione quantomeno opinabile - come si è visto in Aula - abbiano votato come chiesto dal Partito democratico. Sono coincidenze di cui ci limitiamo a prendere atto. La realtà è che questa partita dei Ministri e dei Sottosegretari viene utilizzata dal Partito democratico per sistemare i sommersi e i salvati. si è dimesso positivamente da Sottosegretario; subito dopo è stato nominato Sottosegretario del Governo (per non scendere sotto il livello *record* di 102

Oggi quanto è accaduto - è di tutta evidenza - deriva dalla scelta del Partito democratico di avere un senatore piuttosto che un altro. Il ministro Turco non ha ripresentato le sue dimissioni o, comunque, non sono state poste ai voti.

Nigra - ha aderito al movimento della Sinistra Democratica, quindi, non è conforme all'opinione del Partito democratico. Ebbene, oggi è stato inferto un colpo alla credibilità del Senato e delle istituzioni. Senatore Bobba, l'etica e la questione morale è anche questo, non è solo ciò di cui lei meritoriamente si occupa in altre sedi.

la produzione legislativa, che è il nostro compito. Io ho semplicemente esercitato un diritto di opzione cui la Giunta per le elezioni ha acconsentito; nient'altro. Se non avessi goduto di tale diritto, non sarebbe cambiata la mia vita. Continuo a fare il parlamentare. Non ho altro da dichiarare.

solo dirle, perché con un clima di questo tipo è bene che si conoscano con chiarezza le posizioni di tutti, che per quanto riguarda le decisioni sull'ordine dei lavori di stasera, né io né il senatore Peterlini siamo stati consultati. Non ne faccio una questione, ma è bene, per correttezza dei rapporti e per schiettezza tra di noi, che cambino un po' le modalità di rapporto all'interno del Senato. Presidente, intervengo per precisare che evidentemente ci dev'essere stato qualche disguido nella catena di comunicazione, perché anch'io non sono stato interpellato. Può capitare; evidentemente, la Telecom o Vodafone ogni tanto hanno qualche problema,

dico prima ciò che avrei dovuto dire in conclusione del mio brevissimo intervento e cioè che sono d'accordo con ciò che lei ha proposto poco fa: è di buon senso, è ragionevole. Peraltro, sono d'accordo con ciò che ha affermato il senatore Pera.

Sono lieto di avere interpretato anche il suo pensiero, senatore Cutrufo. Chiaramente è stata mia cura e premura interpellare soprattutto coloro che avevano sollecitato in Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione di queste dimissioni.

per una sorta di accordo trasversale, non è stata fatta propria dal Parlamento europeo, in barba al popolo italiano in nome del quale era stata emessa. Credo

trattandosi di una decisione che dev'essere assunta a maggioranza e non all'unanimità, quando io stesso riscontro, andando personalmente a parlare tra i banchi, un 80-90 credo che a quel punto quelli più in alto potrebbero intervenire per dissentire. Se poi anche loro sono favorevoli, si è fatta una scelta condivisa al 100

apre una nuova finestra") del 23 gennaio 2007, anche in considerazione di quanto accaduto nei giorni scorsi, in merito alla sospensione del giudizio di parificazione del bilancio regionale 2006 della Sardegna da parte della Corte dei conti e l'invio dello stesso alla Corte costituzionale. La Corte dei Conti ha eccepito l'iscrizione di 500 milioni di IVA che sono stati riconosciuti dallo Stato a seguito della vertenza sulle entrate.

si apprestino ad adottare una riforma così rilevante per 945 persone che rappresentano l'intero Paese. Nel momento in cui si sta discutendo di una questione clamorosa, quale l'innalzamento, dal 31 dicembre 2007, di tre anni dell'età pensionabile per tutti i cittadini italiani che hanno oggi 57 anni, io credo sarebbe assolutamente importante, signor Presidente, ferma restando l'assoluta, ovvia e nota competenza del Consiglio di Presidenza del Senato rispetto all'adozione di eventuali provvedimenti di riforma inerenti i vitalizi dei parlamentari,

un essenziale strumento di riforma. Insomma, signor Presidente, non vorremmo trovarci nella condizione nella quale 945 parlamentari si trovano a veder modificata - in un modo o nell'altro, non mi interessa il contenuto, sia chiaro

Mi rendo conto, signor Presidente, che non c'è alcun obbligo in tal senso: sto soltanto facendo appello alla sensibilità nota della Presidenza, in questo momento anche alla sua che la rappresenta totalmente e autorevolmente. È opportuno che quando i parlamentari risponderanno al Paese della propria previdenza, nel momento in cui ci sarà una riforma previdenziale o nel momento in cui scatterà lo «scalone» (il 31 dicembre, se non ci sarà

Ciascuno dei parlamentari, essendo ovviamente una decisione che non viene assunta dall'Aula ma dal Consiglio di Presidenza, ha tra i Segretari, i Vice presidenti e i Questori, una propria delegazione con cui rapportarsi. Mi risulta però, da quanto mi è stato detto dai Questori, che essi hanno preso contatto e hanno informato non solo tutti i membri del Consiglio di Presidenza, ma anche tutti i Capigruppo. Mi auguro che non si sia verificata una situazione come quella precedente:

non so se per decidere definitivamente o meno e sia io che il senatore Lusi abbiamo dunque ritenuto opportuno porre la questione per informare e fare in modo che essi ne abbiano consapevolezza. Ripeto, come ha detto il senatore Lusi, sappiamo che c'è 1'autonomia totale del Consiglio di Presidenza, ma credo che sarebbe un buon costume se almeno sulla proposta operativa, sui contenuti, i Capigruppo fossero informati.

un intervento *ad adiuvandum* sulla proposta del collega Lusi. Penso che, in un momento nel quale il Paese discute in maniera anche preoccupata e tesa del problema della previdenza, sia assolutamente urgente e necessario un intervento sui vitalizi dei parlamentari. Data la delicatezza che è politica, tutta politica, di un tema come questo, credo sia impensabile che il Consiglio di Presidenza, che pure ne ha i pieni poteri, possa deliberare senza un'informazione dettagliata ai senatori su quale sia la determinazione che intende assumere. È troppo forte la valenza politica di questa decisione: sono tra coloro che ritengono si debba decidere in maniera incisiva e credo che dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter difendere la decisione che viene assunta di fronte all'opinione pubblica.

un'omogeneità di comportamento. Perché dico questo? Vorrei che si evitasse - ora e per il futuro - il ripetersi di altri casi Cancrini: è il caso di un deputato